segretario, nel leggerlo, ha fatto correttamente riferimento all'inizio della seduta di ieri mattina quando, per bocca del senatore Eufemi e del presidente del Gruppo di Alleanza Nazionale Matteoli, è stata sollevata la questione delle deleghe del vice ministro Visco, ovvero se tali deleghe fossero state riattribuite allo stesso Vice ministro sulla gestione della Guardia di finanza, in assenza di un provvedimento pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ma in presenza di incontri del vice ministro Visco col nuovo Comandante generale della Guardia di finanza. A quanto abbiamo appreso dal processo verbale (e questi sono documenti particolarmente importanti, un domani chi volesse studiare la storia del Parlamento farebbe riferimento anzitutto ai processi verbali) con indicazione sommaria appare ‑ ma occorre precisare qualcosa di più - che l'opposizione si è limitata a chiedere chiarimenti al Governo e il Presidente del Senato ha risposto non si sa cosa. Vorrei fosse chiaro

Ora, tutto questo non risulta, con il che sembra quasi che l'opposizione si accontenti che il Presidente sia informato senza informare l'Aula. Siccome la vicenda ha riguardato il Senato della Repubblica e il Ministro dell'economia è venuto in oggi possiamo dirlo, Presidente, e perdoni l'espressione apparentemente forte - a mentire sulla sottrazione di deleghe al vice ministro Visco, perché non essendoci stato alcun esercizio di riattribuzione delle stesse non sappiamo cosa è successo al Ministero dell'economia, abbiamo il diritto di sapere immediatamente quali sono le risposte del del Governo al Presidente del Senato. Allora, delle due l'una: o il Governo non risponde, o il Presidente del Senato si rende corresponsabile del silenzio del Governo e questo sarebbe inaccettabile. La preghiamo, quindi, di voler ampliare quel processo verbale perché abbiamo il diritto di sapere che cosa è successo a Via XX settembre.

è sempre una estrema sintesi della discussione che abbiamo fatto e dei quesiti o delle risposte che ad essi vengono date dalla Presidenza. Da un punto vista formale, nel processo verbale non ci sono i dettagli ai quali lei ha fatto riferimento, che però - come giustamente ha ricordato - sono esattamente richiamati - e non poteva essere diversamente

al Governo di avere notizie in merito alla questione sollevata, cioè sulle deleghe al vice ministro Visco conferitegli dal Governo e poi ritirategli secondo l'annuncio del ministro Padoa-Schioppa. Il Presidente del Senato si è attivato presso il Governo per chiedere una sollecita risposta in merito al quesito che era stato posto; posso fare altrettanto

Presidente, colleghi senatori, la mia richiesta di intervento fa riferimento a una questione che oggi campeggia sulle prime pagine di tutti i giornali italiani.

di tutti i giornali italiani. Credo che il Senato della Repubblica abbia il diritto di sapere dal Governo e segnatamente dal Presidente del Consiglio o dal Ministro dell'interno - e per questo, Presidente, mi permetto di avanzarle richiesta di immediata soddisfazione

con l'inquietudine che prende ciascun cittadino di fronte a quanto sta succedendo. La pregherei, Presidente, di prestare un minimo di attenzione ai miei argomenti perché vorrei una risposta precisa. Vorrei sapere

Ci siamo lasciati tristemente alle spalle la vicenda di un generale della Guardia di finanza che è stato definito in quest'Aula «fellone», dopo averlo promosso alla Corte dei conti, salvo poi la sua rinuncia. Questo fa capire che razza di Esecutivo e quali logiche abitano all'interno del Governo Prodi. Arriviamo all'assurdo che nella giornata di ieri, rispondendo ad un *question* *time*, il Presidente del Consiglio fa sapere - e casualità vuole che l'episodio avvenga nello stesso giorno in cui si comunica, qualche settimana o mese dopo, che il dottor De Gennaro è iscritto nel registro degli indagati (guarda la coincidenza con la la risposta all'interrogazione da parte del Presidente del Consiglio) - che sono pronte le valigie per il trasloco dal Viminale del Capo della Polizia, senza dire una parola di più, lasciando allo sbando le forze dell'ordine. Si inventa la favola del mandato settennale. Vorrei sapere da un qualunque membro del Governo in quale norma di legge è scritto che il Capo della Polizia dura in se il Capo della Polizia è efficiente lo si lascia al suo posto finché va in pensione, se invece non funziona non lo si lascia al suo posto un giorno di più. Siamo in presenza di un atto davvero In questo Paese accadono cose strane. Da quello che leggiamo sui giornali, pare che il dottor De Gennaro debba obbedire a un *diktat* dell'estrema sinistra che sostiene il Governo Prodi.

da molti mesi ormai abbiamo presentato un'interrogazione a proposito del Viminale, per sapere se il Ministro dell'interno, anziché accettare la cacciata del Capo della Polizia, non intenda, invece, preoccuparsi di un altro fatto gravemente simbolico all'interno del Viminale, dove un Sottosegretario - guarda caso, anch'egli appartenente ad uno dei partiti dell'estrema sinistra - non ha trovato niente di meglio da fare che assegnare il ruolo di portaborse, di assistente del proprio ufficio ad un terrorista condannato per il delitto Taliercio. Vorremmo che dal Viminale andassero via i terroristi, non il Capo della Polizia! dai Gruppi* *AN e FI)*. Questi argomenti toccano la serenità dei cittadini. Ecco perché vogliamo che il Ministro dell'interno o il Presidente del Consiglio vengano qui a riferire quali sono le intenzioni dell'Esecutivo non fra un anno, non fra un mese, ma oggi,

ma anche al professor Curcio, che tiene lezioni presso le università italiane; subiscono perfino l'oltraggio, pur nel dolore del ricordo della morte di un giovane, di vedere una sala del Senato intitolata ad un estremista che voleva ammazzare un carabiniere.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, come tutti i giornali di oggi riportano, in occasione dello svolgimento della prima prova dell'esame di maturità, si è verificato un errore assai grave, per quanto riguarda il primo tema oggetto di questo esame. Con riferimento, in particolare, alla prova su Dante, ci sarebbe stato uno scambio clamoroso di personaggi e di canti danteschi nell'enunciato della traccia. Ieri sera, è intervenuto sulla vicenda il presidente della Società dantesca italiana parlando di «errore molto grave dovuto a faciloneria» e di «errore fuorviante». Credo che non sia del tutto irrilevante l'ordine con cui i personaggi citati da Dante venivano elencati. È evidente che San Tommaso, San Domenico e San Bonaventura non erano inseriti a caso nei canti

quando è lo Stato stesso a dimostrare una così grave superficialità e incompetenza. Peraltro, credo si tratti di un errore che getta discredito sull'operato dell'amministrazione. Ma questo errore non è un un *unicum*, non rappresenta un fatto isolato. L'altro giorno il vice ministro Bastico assicurava la piena regolarità dell'esame di maturità. Invece proprio ieri abbiamo avuto notizia che ben 400 privatisti qui a Roma non hanno potuto sostenere l'esame. A 400 privatisti è stato negato di sostenere l'esame perché non si era provveduto in tempo utile ad individuare la sede in cui potevano svolgere le prove.

dunque, non provvisti di quella esperienza che si richiederebbe ad un valutatore di un esame così delicato e importante. D'altro canto, il ritardo nella pubblicazione delle commissioni ha comportato anche gravi problemi nella sostituzione dei commissari. So di diverse commissioni che non sono ancora regolarmente costituite. So che esistono commissioni irregolarmente costituite, con commissari non competenti nelle materie in oggetto. dire che sono stati buttati via 150 milioni di euro per riformare la maturità, con risultati che appaiono gravi e deludenti.

da inserire la riforma delle superiori nel decreto dove si parla della rottamazione delle automobili usate. Il ministro Fioroni dovrebbe rispondere con urgenza su questi temi che gettano un'ombra molto grave sulla competenza e serietà del suo Ministero.

Presidente, colleghi, ieri il Presidente del Consiglio, nel rispondere alla Camera ad un atto di sindacato ispettivo, ha comunicato la prossima sostituzione del Capo della polizia,

Questo mi consente due riflessioni, Presidente. La prima: a ben vedere questa norma non scritta è estremamente flessibile, se è vero come è vero che i sette anni scadevano nel mese di maggio, e il Governo non ha ritenuto di procedere alla scadenza di quel termine al cambio del Capo della Polizia.

ma perché oggettivamente siamo d'accordo con quella gran parte del popolo italiano che nelle recenti elezioni amministrative ha, con il voto, dimostrato quanta scarsa fiducia abbia nella attendibilità delle parole del Governo, e in particolare del Presidente del Consiglio. Ma veda, signor Presidente, il problema reale non è forse il cambio del Capo della Polizia, anche se forse correttamente il senatore Pisanu in una intervista rilasciata ieri, e apparsa oggi sulla stampa, mostra alcune perplessità in ordine ad una durata a termine così rigida nei confronti di un uomo delle istituzioni che ha mostrato in questi anni grande capacità nel servire...

molto semplice. Il preannuncio di licenziamento avviene - chissà perché - contestualmente alle notizie concernenti un avviso di garanzia emesso dall'autorità giudiziaria di Genova nei confronti del prefetto De Gennaro - chissà perché - contestualmente alla fuoriuscita di verbali quali, ad esempio, l'esame testimoniale reso dal prefetto De Gennaro nella istruttoria a Genova, che non ci risulta essere allegato al fascicolo del processo.

a noi parlamentari dell'opposizione ma principalmente al Paese, che questo licenziamento è strettamente correlato ai fatti di Genova e, in particolare, ad un avviso di garanzia che sembrerebbe essere stato emesso nei confronti del prefetto De Gennaro. Gravemente, per un verso si utilizza in modo strumentale quell'avviso di garanzia per cercare di trovare quel coraggio che in una situazione normale si è dimostrato di non avere. In secondo luogo, gravemente si consente all'autorità giudiziaria di scandire i tempi della politica e, attraverso i propri atti, di decidere del destino degli uomini. Presidente, non è serio ed è davvero molto distante da quella serietà che il presidente Prodi assume essere

occorrerebbe non farsi prendere la mano - mi permetta, senatore Storace - dalla propaganda strumentale e trattare la questione con grande correttezza. Credo che ieri il Governo, attraverso le parole del Presidente del Consiglio, abbia agito correttamente.

Nessuna destra ha mai oltrepassato un limite, che è sacro, che è dentro il contratto sociale, direbbe Rousseau, che è dentro il contratto di convivenza democratica. Non si tenta mai da parte dell'opposizione di schierare le forze dell'ordine e militari contro il Governo e la maggioranza parlamentare, nonostante l'autonomia della critica, laddove questa sfiducia può ingenerare anche una inquietante presa di distanza fra politica e poteri militari. *(Commenti del senatore Storace).* È la nostra Costituzione che dice che il potere politico non è ancella, non è serva del potere militare. Non vogliamo una politica serva. Non dubitiamo - lo ripeto per l'ennesima volta - della legalità democratica e costituzionale delle forze dell'ordine. Il tema centrale non è l'essere a favore o contro le forze dell'ordine. Sarebbe un venir meno ai propri diritti e doveri di parlamentari. Il tema, invece, è la centralità della Costituzione, del giuramento sulla legalità costituzionale. Sono stato otto anni

perché delle torture a Bolzaneto - e crediamo di averlo dimostrato - perché la Diaz, perché la macelleria messicana, come ha detto il vice questore Fournier. Noi non attacchiamo, senatore Storace, le forze dell'ordine; non facciamo propaganda; non difendiamo i *black bloc*, come lei ha detto per televisione. Noi crediamo che l'onore ed il rispetto delle forze dell'ordine siano rafforzati da un'inchiesta seria su quello che non solo il vice prefetto**,** ma chiunque conosce le forze di polizia

Pregherei i colleghi che devono intervenire - lo hanno chiesto a norma del Regolamento e, ovviamente, non posso non dare loro la parola, rispettando io stesso per primo il Regolamento alla lettera - di attenersi alle questioni che intendono sollevare. Il rischio è di una discussione che tracimi nel merito di una vicenda che ancora mi sembra tutta aperta, discussione che noi facciamo impropriamente, tra l'altro senza la presenza del Governo, come era stata sollecitata nell'intervento primo del collega Storace.

Non credo che il primo che chiede la parola stabilisca, in qualche modo, l'ordine del giorno. Siccome vorrei richiamare una questione analoga, credo di avere il diritto di poterlo fare come i colleghi che sono intervenuti sulla questione del Capo della Polizia (su cui dirò qualche parola alla fine).

Presidente, già sussistevano dubbi sulla legittimità dell'affidamento di quella delega, perché l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189,

Quanto invece alla questione del Capo della Polizia vorrei dire solo due parole, Presidente. Non condivido alcune delle considerazioni fatte dai miei colleghi dell'opposizione e, a differenza loro, ritengo che il Governo abbia fatto bene a rimuovere il Capo della Polizia. Su di lui il mio giudizio coincide con quello espresso in quest'Aula dal presidente Cossiga in alcuni suoi atti ispettivi. Ai miei colleghi voglio far presente che se quanto ha detto l'onorevole Russo Spena fosse effettivamente accaduto, e ancora non lo sappiamo con certezza di prova, ciò sarebbe accaduto

è stata annunciata la sostituzione del Capo della Polizia con una motivazione formale che effettivamente non convince nessuno.

lo sostiene ma poi ne chiede la sostituzione) si aggiunge l'altro episodio del generale Speciale della Guardia di finanza. finanza. I due fatti insieme aggravano la situazione e ci fanno dire che c'è sicuramente un problema di rapporto tra il Governo, le Forze armate e le forze dell'ordine.

inoltre della debolezza del Governo e, per altro verso, dell'arroganza di questa maggioranza, che pensa di fare tutto quel che vuole e di sostituire anche in questo settore, come ha fatto in tutti gli altri, i vertici dell'amministrazione.

alla Presidenza qualche valutazione sulla circostanza che stiamo di fatto imponendo una nuova prassi: all'inizio di ogni seduta c'è un'ora, più o meno, di dibattito sull'argomento che il primo che si alza sceglie. Bisognerebbe a questo punto formalizzare la procedura, per impedire che i lavori del Senato vengano travolti da tale prassi. Non sto discutendo dell'argomento in auge questa mattina, perché la prossima mattina ce ne sarà un altro. Prendiamo atto che dopo un voto, con verifica del numero legale, sul verbale della seduta precedente, il Senato ha bisogno -

il fatto che i lavori del Senato non abbiano, come ha detto poco fa il collega Morando, uno svolgimento coerente nel momento in cui vi sono delle emergenze e delle discussioni che originano di giorno in giorno a seconda dei temi sul tappeto. Voglio auspicare

per analizzare i temi più urgenti che sono sul tappeto quanto quella di sentire il Governo anche al Senato in relazione alle questioni che il presidente del Consiglio Prodi ieri ha esposto alla Camera dei deputati sulla futura sostituzione, o destituzione morale, del prefetto De Gennaro. È comunque fuor di dubbio che il Governo e la maggioranza danno spazio quasi quotidianamente ad osservazioni di carattere politico non di poco rilievo.

i fatti del G8 di Genova, e come solo un paio di settimane fa abbiamo discusso la destituzione del generale Speciale della Guardia di finanza. È evidente, credo, che l'approccio del Governo alle sostituzioni, o destituzioni, di importanti cariche dello Stato (il comandante generale della Guardia di finanza il comandante della Polizia di Stato) lasciano spazio a grossi dubbi di carattere politico-istituzionale, diciamo di opportunità, anche se forse bisognerebbe dire di più. È gravissimo, in poche parole

ma vi sono questioni politiche che hanno avuto la loro rilevanza nel tempo passato e che dicono quanto sia effettivamente vero e confermato che la maggioranza e il Governo vogliono sostituire De Gennaro - la cui condanna probabilmente era già segnata il giorno in cui voi del - sotto il ricatto della sinistra estrema e massimalista che vuole fare pagare a De Gennaro e ad altri funzionari di polizia gli eventi del G8 del 2001,

spiegazioni al Governo circa l'eventuale avvicendamento al vertice del Dipartimento di pubblica sicurezza di cui si è parlato legittimo che chieda spiegazioni, legittimo che ponga la questione in quest'Aula, chiedendo alla Presidenza di interpellare il Governo e di concordare un'occasione di confronto. Detto questo, signor Presidente, cari colleghi, il dibattito che si è aperto rischia di essere fuori luogo e fuorviante.

Può esistere una regola di opportunità, che è stata enunciata in questi mesi da fonti responsabili, secondo la quale sarebbe bene che un funzionario che occupa posizioni di vertice così rilevanti non superi

ad offrire o a negare - ed entrambe le scelte sarebbero istituzionalmente sbagliate - una sponsorizzazione politica ad un funzionario che svolge una funzione così delicata

che dirige il Dipartimento di pubblica sicurezza, nel momento in cui esercita le sue funzioni ha in ogni attimo

in un'istituzione così importante. Certo, è possibile che vi sia. È anche possibile che, come già è avvenuto quando abbiamo al tempo io stesso avevo la delega relativa alla Polizia di Stato e quindi ho seguito da vicino quella procedura - il Governo consulti l'opposizione o manifesti all'opposizione le proprie intenzioni. Una scelta sul terreno dell'opportunità, del *fair play* istituzionale, che non è dettata naturalmente da nessuna norma e che non stabilisce alcun precedente, ma che, tuttavia, può essere compiuta, come anche noi facemmo nel 2000.

che il Governo potrà manifestare le proprie intenzioni e rispondere alle richieste che sono state avanzate dall'opposizione. Vorrei dire ai colleghi dell'opposizione: dopo le polemiche delle scorse settimane, fermiamoci; garantiamo insieme, perché questo è un impegno comune, l'imparzialità necessaria dei funzionari che svolgono attività così delicate ed anche la loro tranquillità, al di fuori della polemica politica.

è stata manifestata da esponenti della maggioranza e non necessariamente dalla sinistra radicale. Ricordo che il primo ad avere posto il tema è stato l'onorevole Villetti, capogruppo dello SDI alla Camera, che ha posto un problema di responsabilità oggettiva che esiste. È evidente che a Genova è accaduto qualcosa di molto grave che in una democrazia non può essere accettato impunemente. Un alto funzionario dello Stato, che merita anch'egli rispetto e attenzione, ha parlato di macelleria messicana. A tutti sono note le immagini di quello che è accaduto nella scuola Diaz, a Bolzaneto e così via. Credo che esista un principio di responsabilità oggettiva che dovrebbe essere fatto valere più spesso per i politici, ma non solo per essi. Delegare, infatti, tutto alla magistratura penale è un limite di un sistema politico debole. Credo, quindi, che sia giusto che si proceda alla sostituzione del Capo della Polizia perché - ripeto - in una democrazia, se accadono cose estremamente gravi come sono accadute a Genova (e se ci sarà la Commissione d'inchiesta si avrà modo di approfondire, anche se mi pare del tutto evidente che è accaduto qualcosa di molto grave a danno di giovani ragazzi inermi che avevano manifestato, come avevano il diritto di fare, contro il G8), è giusto che chi ha il controllo delle operazioni di polizia ne debba rispondere oggettivamente. Quindi, dal nostro punto di vista è giusto che, alla luce delle risultanze emerse, si proceda in tempi rapidi alla sostituzione del Capo della Polizia.

per il rischio di creare situazioni nuove o, comunque, giammai determinate in quest'Aula. Credo sia esattamente il contrario, atteso che (il collega Morando lo ricorderà) anche nelle passate legislature si dava questa possibilità e a me sembra un fatto corretto. Del resto, anche per quanto abbiamo sentito di fronte al tema posto dal collega Storace, di un'occasione per riflettere su quelle gravità che quotidianamente in qualche modo coinvolgono la politica. Quindi io lo saluto come un fatto positivo, signor Presidente, e mi auguro invece che possa trovare anche un riflesso nel Regolamento, in modo organizzato, onde evitare che il Palazzo sia lontano dalla Nazione per fatti gravi ed importanti che pure accadono nel Paese. MORANDO

così dire, che sarebbero stati commessi dal Ministero della pubblica istruzione nel definire la traccia del tema d'italiano che è stato dato ieri all'inizio degli esami di maturità e che si riferivano specificatamente a Dante e ad una citazione

giunti i testi, le tracce su cui avrebbero dovuto svolgere la prova di italiano. Anche su tale questione abbiamo chiesto al Governo di intervenire.

sul problema molto delicato dell'avvicendamento del Capo della Polizia che, soprattutto dopo quello del generale Speciale al comando della Guardia di finanza, trova particolarmente sensibile sia l'opinione pubblica che il Parlamento. Penso sia giusto e corretto che affrontiamo questo tema per restituire serenità ai cittadini nel rapporto tra Governo, istituzioni e e società italiana. Credo anche che dovremmo affrontare questioni così delicate, come quelle dell'avvicendamento di un Capo della Polizia o di un generale dei Carabinieri o di un capo della Guardia di finanza avendo ben presente la necessità di tutelare i Corpi di polizia e i Corpi militari, in questo caso tutelando la Polizia di Stato e i suoi uomini.

mi preme sottolineare ai colleghi che il tema è stato posto dal Presidente del Consiglio intervenendo nel *question time* ieri alla Camera dei deputati. Il Presidente del Consiglio ha detto (lo riferisco per semplice informazione ai colleghi): «l'opera del capo della polizia è riconosciuta sia in ambito nazionale, sia internazionale. Quanto alla durata del suo mandato, devo riferire che lo stesso dottor De Gennaro lo aveva messo a disposizione contemporaneamente alla nascita del mio Governo. Quando fece ciò, in risposta e a conferma della nostra fiducia, il Ministro dell'interno, il sottoscritto e il dottor De Gennaro avevamo convenuto che, alla scadenza del settimo anno di incarico,» (quindi era una convenzione

In seguito a questa dichiarazione, che è stata resa nota ieri alla Camera dei deputati, si è avuta notizia di una iniziativa della magistratura

che è oggetto dell'inchiesta della magistratura, difendere il Corpo della Polizia di Stato e contemporaneamente difendere le prerogative del Parlamento, insieme però anche a quelle del Governo. Credo quindi sia giusto che il Governo venga a riferire in Senato come è stato chiesto. Infine, è stata sollevata una questione di carattere regolamentare dal collega Morando, in sostanza ha detto che si è qui introdotta una prassi secondo la quale un'ora dell'inizio delle nostre sedute viene praticamente, o costantemente o assai frequentemente, dedicata alla segnalazione di varie questioni e di vari problemi che emergono nel dibattito tra politica e istituzioni, tra società civile e istituzioni, o per effetto di inchieste della magistratura, o magari per effetto di pubblicazione di notizie particolarmente rilevanti che si riferiscono a registrazioni di telefonate o a pubblicazioni di verbali di interrogatori della magistratura su diverse questioni. Di alcune di queste questioni, però, senatore Morando, mi faccia dire, la rilevanza è tale che onestamente credo sia giusto e doveroso che si intervenga doveroso che si intervenga e mi meraviglierebbe il contrario, se i parlamentari non intervenissero, perché in tal caso saremmo in presenza di una sorta di sordità del Parlamento a ciò che gli accade attorno. Possiamo convenire che in sede di Conferenza dei Capigruppo si stabilisca che 40‑45 minuti vengano in questo senso dedicati alla segnalazione dei problemi.

Non è prassi di questa Presidenza né compiere qualcosa di illegittimo, né rendersi complice di qualcosa di illegittimo, ma soltanto ed esclusivamente questa Presidenza si attiene all'applicazione rigorosa della lettera e del dettato del Regolamento del Senato della Repubblica.

dei senatori Storace e Valditara, hanno partecipato al dibattito con molto senso di responsabilità: non lo condivido, ma mi riferisco in modo particolare all'intervento molto sereno e appropriato però qui denunciare un aspetto. Lei,signor Presidente, molto abilmente ha risposto, ma ha svolto due ruoli: quello di Presidente del Senato

per sapere se si possono avere notizie sull'incendio che ha colpito il policlinico Umberto I di Roma, dove il quarto padiglione - sembrerebbe per un corto circuito - è andato completamente distrutto. In questo momento si stanno evacuando

negli interventi che il Governo si è impegnato ad introdurre nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Mi limiterò quindi a due ordini di osservazioni nel merito delle questioni connesse alla discussione di questo disegno di legge. al richiamo che, in materia di tutela della salute e di sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, è stato fatto alle lotte del movimento operaio e dei movimenti politici delle donne. delle donne. In quest'Aula si è parlato appunto di soggetti che sono socialmente, ma anche sessualmente, connotati e si è detto che non è soltanto una questione di condizione, ma è soprattutto una questione di soggettività politica, di capacità di produrre cultura politica e un'idea di una società diversa. In sostanza, parlo della trasformazione dei rapporti sociali che definire incivili è - credo - un eufemismo di fronte alla drammaticità dei dati che ci sono stati ricordati.

e quando furono modificate le catene di montaggio per rendere loro possibile l'accesso al lavoro. Lì si realizzò un principio fondamentale che oggi è stato pesantemente rimesso in discussione: quello, cioè, che un processo produttivo deve essere a misura del lavoratore e della lavoratrice e non questi ultimi a misura del processo produttivo, processo produttivo che oggi esce dalla fabbrica. Credo che il movimento per il superamento dell'*handicap* ci abbia anche consegnato, attraverso la legge n. 104 del 1992 (una legge molto importante, capace di rileggere il diritto alla salute come diritto trasversale, che taglia tutti gli altri

il quale dovremo confrontarci nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Ma soprattutto - e questa è la seconda riflessione che vi sottopongo la stessa legge n. 104 del 1992 ci rinvia, così come la nuova Convenzione dell'ONU per i diritti umani delle persone con disabilità, a quell'idea fondamentale su cui si fonda l'articolo 32 della Costituzione, cioè al ruolo che spetta alla salute in termini di diritti umani; non solo quindi il suo mantenimento e il suo recupero sono un bisogno un bisogno riconosciuto come diritto e una risorsa fondamentale per l'individuo, per la sua libertà e per la sua realizzazione, ma sono soprattutto un interesse di questa società. Lo sono, quindi, la salute delle lavoratrici e dei lavoratori e lo sono non solo nei luoghi di lavoro. Credo che questa presa di coscienza, che è patrimonio comune di tutti i movimenti di lotta che qui ho richiamato, riguardi anche le disuguaglianze nella salute, che contraddicono quelle aspettative che nel 1978 alla Conferenza di Alma Ata aveva fatto generare l'obiettivo della salute per tutte e tutti nel 2000 (parlo del nostro Paese, ma c'è anche un problema di relazioni con altri Paesi, con i Paesi cosiddetti del Terzo mondo). Quell'obiettivo non solo non è stato raggiunto, ma le disuguaglianze nella salute, collegate in particolare alla condizione del lavoro subordinato,

C'è un livello di povertà collegato, appunto, alla questione salariale, alla drammatica precarizzazione dei processi di lavoro e alla perdita reale di potere d'acquisto delle pensioni in questo Paese. Abbiamo i salari e le pensioni più bassi d'Europa

euro. Questo dato ci parla anche dell'equità nell'accesso ai servizi sanitari, sia a quelli di prevenzione che a quelli di diagnosi e cura. Abbiamo svolto in Commissione sanità un'indagine conoscitiva sulla libera professione medica intramuraria in relazione all'equità nell'accesso e abbiamo preso atto che molti dei servizi di specialistica e diagnostica sono solo teorici e che le prestazioni, persino quelle urgenti, rese nel Servizio sanitario nazionale vengono prestate in tempi superiori a quelli nei quali si può ottenerle attraverso la libera professione intramuraria dei medici, cioè con costi che arrivano ai 1.000 euro e che mediamente si aggirano sui 250-300 euro. euro. Questo dato, correlato con le difficoltà del 30 per cento delle famiglie italiane, ci parla della necessità di un intervento che ristabilisca l'equità e che rimetta le famiglie, le donne e gli uomini

Quindi, abbiamo un problema anche di casa, di affitti che si mangiano stipendi e salari, e abbiamo un problema in relazione alla non autosufficienza e alla carenza dei servizi;

che si chiamava Giorgio La Pira, il quale nel 1978, quando gli si chiese perché sosteneva la necessità di un Servizio sanitario a carattere universalistico finanziato sulla fiscalità generale, rispose: sì, io voglio pagare la sanità per Agnelli perché finché sarò curato nello stesso ospedale dove si cura Agnelli sarò sicuro che non ci saranno diseguaglianze tra la sua salute e la mia.

credo che questo provvedimento non evochi un crescendo di attenzione e, quindi, anche di definizione Prego i colleghi del Gruppo dell'Ulivo di sciogliere quell'assembramento. Mi riferisco al senatore Antonio Boccia, al senatore Goffredo Bettini e agli altri.

in Commissione - dobbiamo dirlo - serenamente, senza alcun elemento precettivo. Di fatto, conteneva

insieme al presidente della Commissione lavoro, il senatore Treu,

propri di una dialettica tra maggioranza e opposizione che, a nostro avviso e ad avviso della maggioranza, non potevano trovare albergo in un tema così importante e da tutti fortemente sentito. sentito. Il lavoro della Commissione ha prodotto una serie di norme immediatamente esecutive, dopo l'approvazione definitiva del disegno di legge, ed in parte ha riequilibrato ciò che doveva essere una delega generale introducendo una serie di norme precettive.

creare in questo ramo del Parlamento una Commissione di inchiesta sul fenomeno, il Governo non può non tener presente tutto ciò.

copertura, si prendano tre punti percentuali del tesoretto per dare una copertura che permetterà ulteriori norme precettive che accompagneranno la definitiva approvazione del disegno di legge sia alla Camera che al Senato.

lo Stato rimette nel Piano sanitario cifre che riguardano anche la destinazione mirata alla prevenzione in modo complessivo.

Non ci si può assolutamente nascondere dietro procedure o consuetudini o, addirittura, tavoli che spesso non producono atti. Bisogna osare. Bisogna dare risposte concrete. Bisogna attenzionare veramente questo tema, altrimenti si rischia di essere sempre sensibili, si rischia che ogni volta che accade un dramma il tutto si consumi in poche ore, con una serie di esternazioni di solidarietà o di condoglianze nei confronti delle famiglie e delle persone che hanno perso un loro congiunto vittima di un infortunio sul lavoro. Non credo che

(molti sono rappresentati dal relatore e dal Presidente di Commissione), ci vedono convergere. Sono - se mi posso permettere, presidente Treu, collega Roilo - emendamenti condivisi da tutti, quali è stato detto che avremmo trovato in Aula il necessario supporto e la necessaria copertura economica. Ebbene, non solo non li si trova in Aula, ma addirittura si vuole tagliare su quei temi che già erano stati oggetto di voto favorevole da parte della Commissione. Mi riferisco, ad esempio, al credito di imposta, che si vuole ridurre da una copertura di 25, che pure era stata data, a 10 milioni;

della materia relativa al tema della sicurezza del lavoro in ogni percorso di formazione professionale e nei programmi scolastici ed universitari.

e dell'organizzazione (propria del Ministero, al quale fanno riferimento questi organi di istruzione), di insegnamento di insegnamento della cultura del lavoro, per fare in modo che questo tema possa in prospettiva essere compreso; esso deve essere sicuramente oggetto di riflessione e approfondimento già dalle scuole elementari

cui saranno necessarie precauzioni al fine di evitare incidenti, infortuni e drammatiche morti. Di fronte a tutto ciò, mi auguro che il Governo voglia ritirare gli emendamenti che riducono e vanificano - di questo mi dispiace - il tanto lavoro svolto in Commissione

Ci è stato detto che bisognava aspettare il 20 giugno per la relazione semestrale di cassa. Ci siamo arrivati. arrivati. Anche da questo punto di vista il Governo ha tutti gli elementi per valutare se intende licenziare un testo che dia risposte concrete concrete e che sia in linea con le attenzioni delle massime autorità dello Stato, oppure se vuole licenziare un testo di basso profilo, che credo nessuno all'interno di quest'Aula riesca a condividere ed accettare.

sin dall'inizio della discussione del provvedimento abbiamo provveduto a regolare la nostra posizione ritirando financo le questioni pregiudiziali che erano state presentate, perché abbiamo pensato che il provvedimento stesso non potesse essere considerato per quello che veniva percepito all'esterno e quindi assolutamente necessario. giusto dibattito nel Paese e nelle Aule parlamentari da tempo coinvolge le rappresentanze sia dei lavoratori, sia delle

a tutela della sicurezza dei lavoratori. Veniva però rilevato dalla nostra parte politica e dai senatori che più di me si sono occupati della vicenda, come l'ex sottosegretario Sacconi e il collega Morra, Morra, che il provvedimento aveva una specifica e carente copertura finanziaria. Cioè, non erano specificati gli oneri, non erano specificati gli oneri, in special modo con riferimento a quelle misure aggiuntive che si prevedeva dovessero essere adottate dalle amministrazioni pubbliche e dai datori di lavoro,

un ampliamento ulteriore rispetto alle vigenze legislative. Ciò è stato fatto altre volte; si dirà che comunque i testi dovranno essere presentati alle Commissioni competenti per il parere. Ma il parere finisce, come sappiamo benissimo, per essere consultivo, per non essere determinante. La nostra preoccupazione è stata pertanto che si potesse configurare

più cogenti e più pressanti, che non accompagnavano la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro e quindi facendo sì che certi sistemi di tutela venissero introdotti

Ma cosa c'è ancor di più? Come fare a non essere d'accordo a migliorare la sicurezza sul lavoro? Come fare a non essere d'accordo con le teorie di Taylor, riprese dal dal francese Fayol e poi rivisitate in tutta la moderna teoria sull'organizzazione del lavoro? Come non considerare che ciò di cui oggi discutiamo non è certamente riconducibile a fattori motivazionali nel mondo del lavoro, ma soltanto a fattori igienici? La sicurezza sul lavoro è, cioè, il principale

sia totale. Noi non siamo stati ostativi; credo siamo fortemente positivi, siamo prudenti nella manifestazione della nostra posizione, ma riteniamo che tutto questo non sia consentito dalla delega

in Commissione, in special modo nella 5a Commissione (bilancio e programmazione economica), è che i criteri di delega che vengono descritti all'articolo 1 del provvedimento in esame

la definizione del quadro finanziario, la quantificazione degli oneri e la relativa copertura devono essere effettuati in sede di legge di delega e non rimandati ai decreti legislativi. Tutto ciò non è presente

È un fatto positivo - hanno detto altri colleghi - che, oltre all'articolo 1 e oltre ai criteri di delega, vengano assommati tanti altri articoli che arricchiscono la legislazione che deve essere presa a riferimento della legge delega per

mentre è chiaro che la sicurezza sul lavoro non può che essere considerata un fattore igienico e non motivazionale, tale impostazione viene travolta e stravolta dai fondamenti ideologici e prodromici della sinistra più più estrema della maggioranza, che tende a contrapporre il perseguimento della sicurezza del lavoratore al giusto interesse del datore di lavoro.

E se è la ricchezza della stessa azienda, la sanzione nei confronti del datore di lavoro non può essere quella richiamata nelle disposizioni aggiuntive a questo testo. Siamo d'accordo sul fatto che debba essere svolta più formazione, sul fatto che si proceda all'assunzione di quegli ispettori del lavoro, la cui prima parte era stata già chiamata in servizio nella precedente legislatura, ma non siamo d'accordo con questa attività attività legislativa assolutamente persecutoria di un mondo del lavoro che, dove coniuga nell'impresa il lavoro e il capitale,

e il diniego dei diritti igienici del lavoratore. Allora, proprio per questo, come diceva poc'anzi il senatore Tofani, non comprendiamo la scarsa attenzione del Governo all'individuazione delle giuste

non dà quella risposta che l'opposizione, con un'attività di enorme e fattiva collaborazione in Commissione e in Aula, sta richiedendo per fare sì che questo provvedimento sia di giusta risposta non ad una pretesa, ma ad un'attesa che tutta la popolazione italiana ha sopportato, sensibilizzata specialmente dagli orrendi fatti e dalle disgrazie avvenute di recente nel mondo del lavoro. Non è pensabile che l'obiettivo venga venga perseguito attraverso un provvedimento che è contraddittorio tra il primo articolo e gli articoli che rinnovano, aggiungono, novellano

alle risorse previste nella finanziaria al comma 780, dove si dice specificatamente che quelle erano risorse originate da un tasso d'incremento del gettito contributivo complessivo relativo e, comunque, e, comunque, per un importo non superiore a 300.000 euro. Ma quelle erano risorse evenienti e non delle risorse certe, tanto che proprio in Commissione bilancio si è dovuta porre una condizione, ricevuta nel testo, che

attività di promozione della cultura e delle azioni di prevenzione da finanziare non potranno che aver luogo che a decorrere dall'esercizio 2008 e che potranno essere

tiene conto di una letteratura che è stata assolutamente e totalmente rinnovata, dicevo poc'anzi, non soltanto da Fayol rispetto all'atteggiamento terroristico dello dello sfruttamento - se una volta soltanto e soltanto una volta si vuole richiamare questa orrenda parola - ma anche rispetto alla relazione tra datore di lavoro e prestatore d'opera, che non esiste più in quella filosofia che è richiamata dalla sinistra estrema della maggioranza.

pericolosa penalità che si vuole introdurre nei confronti del datore di lavoro. Oggi non ha significato e trova testimonianza in un atteggiamento retrivo della sinistra e della maggioranza che riteniamo non possa e non debba essere introdotto in quel testo unico, per cui

sottolineare i punti positivi e i progressi che abbiamo insieme ottenuto, rispondendo magari a qualche critica forzata.

Qui ci si muove molto sul piano dell'effettività, quindi occorrono organizzazione, intervento pubblico, controllo sociale. Qualcosa è stato fatto, perché i provvedimenti iniziali che

di estenderla tenendo conto delle specificità, dei rischi particolari e delle condizioni, anche secondo - come abbiamo scritto - le indicazioni dell'Unione Europea. Sottolineo anche l'allargamento dell'ambito applicativo molto importante, i nessi tra sicurezza interna ai luoghi di lavoro e le conseguenze sull'ambiente esterno; poi, tutta la grande area degli appalti, dei subappalti, delle catene di esternalizzazione che, se non controllate, creano le occasioni più gravi di infortunistica. Anche su questo abbiamo

ad alcuni punti che sono stati rilevati anche con qualche critica - ripeto - forzata, ma che invece una parte dell'opposizione ha concordato. Anzitutto, la semplificazione,

indicazioni precise, alcune di delega, altre con effetto immediato: ad esempio, abbiamo indicato l'obiettivo dell'unificazione documentale che è importantissimo

fondamentali per la prevenzione: abbiamo introdotto un rafforzamento delle rappresentanze sindacali ai vari livelli, che sono uno strumento anche di prevenzione e per questo abbiamo previsto della formazione specifica; abbiamo introdotto rafforzato le tecniche di monitoraggio; abbiamo previsto un obbligo di formazione per la qualificazione delle imprese che va nella medesima direzione; abbiamo accolto anche indicazioni dell'opposizione sul cosiddetto interpello, che serve a questo,

interventi per obiettivi si può accettare in senso lato, ma non è che siamo in una normativa, come quella per esempio del mercato del lavoro, per cui si indica un obiettivo importa come lo si raggiunge, qualcuno può fare una cosa, qualcuno ne può fare un'altra. Gli obiettivi sono importanti, ma trattandosi di normativa che ha a che fare con la salute e la sicurezza dei lavoratori alcune norme rigide ed imperative

è stato discusso a lungo. Vi sono critiche all'attuale impianto un po' da tutte le parti. Per qualcuno siamo troppo repressivi, per qualcun altro saremmo stati assolutori. Credo piuttosto che abbiamo

Abbiamo richiesto, inoltre, di graduare le sanzioni per certi soggetti particolarmente esposti, come i cosiddetti preposti. Abbiamo previsto normative sanzionatorie, come le pene interdittive, per i casi gravi. Ma abbiamo dosato nella convinzione che si debba valorizzare il cosiddetto ravvedimento e che si debba accompagnare alla sanzione anche l'incentivazione e il premio per i comportamenti virtuosi. Per questo motivo, abbiamo valorizzato le buone prassi.

abbiamo condiviso molte di queste norme e abbiamo ritenuto che su alcuni punti - in particolare sulle norme immediatamente precettive - si debbano

Signor Presidente, anch'io ho apprezzato - lo dico senza nessun atteggiamento formale - il dibattito molto impegnato che si è svolto in Aula, così come

non c'è tutta questa urgenza di procedere sul piano normativo, anche perché il fenomeno degli infortuni sul lavoro è in calo.

Inoltre, il livello attuale è praticamente stabile da diversi anni e si trova stabilmente al di sopra delle mille unità.

di norme tendenti principalmente a riordinare la materia e ad adeguare le normative del nostro Paese a quelle europee. Oggi abbiamo un testo

e si fonda su due pilastri: la prevenzione da un lato, con la diffusione della cultura della sicurezza e delle buone prassi, le misure premiali soprattutto per le piccole e medie imprese, la formazione, la qualificazione delle imprese, meccanismi per stabilire l'idoneità tecnico-professionale delle imprese ai fini della partecipazione agli appalti pubblici, l'integrazione dei sistemi informativi, il potenziamento degli organismi paritetici, il coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza, i controlli, con il coordinamento della vigilanza, l'incremento del personale ispettivo, la sospensione delle attività per gravi e reiterate violazioni della normativa sulla sicurezza, l'interdizione all'accesso di benefici di finanza pubblica per le imprese non virtuose. Infine, le sanzioni che sono equilibrate e che rappresentano non una formalistica adesione ad un intento punitivo nei confronti dell'azienda, ma un deterrente serio perché calibrate sulla gravità delle infrazioni. previsto un inasprimento di esse, proprio come deterrente efficace. Tale inasprimento si accompagna all'implementazione del catalogo dei reati presupposto per l'affermazione delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche, estendendolo all'ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose commesse in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. lavoro. Ciò consapevoli dell'esigenza di un sistema sanzionatorio misto che combini l'impiego delle sanzioni di diversa natura. I princìpi cardine del testo della delega, contenuti all'articolo 1, sono rappresentati, come poc'anzi è stato ricordato dal senatore Treu, dall'estensione del campo di applicazione. La Commissione lavoro ha, inoltre, integrato l'articolo 1 migliorandolo anche con riguardo alle differenze di genere e alle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Altro principio fondamentale è rappresentato dalla garanzia della uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale finalizzato ad evitare diversificazioni in una materia che riguarda beni fondamentali per la persona, come la salute e la sicurezza sul lavoro. Mi preme sottolineare che tale esigenza, oltre ad essere stata più volte rimarcata nel dibattito svolto in Commissione, è stata condivisa anche dalle Regioni attraverso il parere favorevole espresso sul disegno di legge delega dalla Conferenza Stato-Regioni. Ne deriva che allo Stato spetterà individuare nel decreto di attuazione i principi generali sui minimi delle tutele che costituiranno un nucleo intangibile rispetto al quale la potestà legislativa concorrente delle Regioni potrà realizzare deleghe migliorative esercitando le proprie competenze. Ascoltando anche i rilievi della Commissione lavoro e la richiesta avanzata dalla Commissione d'inchiesta sugli infortuni, oltre che quelli delle parti sociali, abbiamo scelto

in maniera da rispondere alle esigenze più urgenti, in attesa del completamente del disegno di riforma. Tra queste vorrei ricordare la norma sul coordinamento della vigilanza affidata ai Comitati regionali di coordinamento che riteniamo di fondamentale importanza, quella sull'integrazione degli archivi informativi da parte degli enti e delle amministrazioni con competenze in materia e l'avvio di progetti sperimentali, già nell'anno scolastico 2007-2008, in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. L'esame del provvedimento da parte della Commissione lavoro ha poi consentito di introdurre nuove norme che hanno reso il testo più completo. Tra queste vorrei ricordare: il riconoscimento alle organizzazioni sindacali e all'associazione dei familiari delle vittime, della possibilità di costituirsi in giudizio, la revisione dei requisiti e delle funzioni del medico competente, la previsione della specifica indicazione nei bandi di gara per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture dei costi della sicurezza, l'introduzione dello strumento dell'interpello, la tessera di riconoscimento per il personale dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice, l'esclusione dei costi della sicurezza

1198 della finanziaria che esclude dalla sospensione delle ispezioni, per le aziende che hanno presentato istanza di regolarizzazione, quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

la normativa che riguardava l'assunzione degli ispettori, che è stata approvata in Commissione nonostante alcune perplessità manifestate dal sottoscritto, presentava una assunzione per circa 600 lavoratori, ossia tutti gli idonei. L'organico del Ministero del lavoro - l'ho fatto presente - è di 400 lavoratori. La copertura finanziaria era limitata soltanto agli stipendi e non alle spese per l'attività, ai buoni pasto e alle spese di missione, ed essa, seppure formalmente ineccepibile,

le istituzioni scolastiche determinano nel piano dell'offerta formativa il *curriculum* obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Le tematiche in questione, comunque, saranno recepite nell'indicazione nazionale per il primo ciclo attualmente in fase di revisione, come saranno oggetto di particolare attenzione in sede di definizione delle linee programmatiche relative al secondo ciclo. Quindi, si rileva una adesione completa alla volontà

sicurezza debba rappresentare un terreno comune di dialogo tra le istituzioni, le forze politiche e sociali, sul quale realizzare quel serrato confronto e quella ricerca di convergenze di cui il mondo del lavoro e l'intero Paese hanno urgente bisogno. Credo che dovremo continuare a lavorare con questo

debbano essere garantiti in ogni caso. Faccio l'esempio dell'obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi,

interviene sui criteri volti a stabilire la composizione numerica delle figure professionali nelle Aziende sanitarie

Signor Presidente, i nostri emendamenti sono coerenti con i rilievi che abbiamo rivolto a questo provvedimento nel corso della discussione generale. In primo luogo, un emendamento ha lo scopo di garantire maggiore tempestività all'entrata in vigore del decreto delegato che dovrà essere prodotto, in base a questo disegno di legge delega, sulla base della conclamata esigenza di garantire quanto prima un Testo unico per dare certezza ed effettività alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nel lavoro. Ed, invero, ci sembra che nove mesi, tempo idoneo per altri profili fisiologici, non lo siano altrettanto per la produzione di un decreto delegato, che sarà redatto sul solco di un'ampia elaborazione che negli ultimi dieci anni è stata intensamente prodotta. In secondo luogo, alcuni emendamenti sono rivolti a garantire risorse adeguate agli obiettivi, anche in questo caso da tutti riconosciuti, di maggiore investimento nella prevenzione, nell'informazione e nella formazione. In modo specifico proponiamo che l'INAIL, sulla base dell'esperienza già realizzata, possa disporre di un fondo che ripete l'attività di finanziamento che l'istituto in passato ha ha svolto nei confronti di quelle piccole imprese che realizzano investimenti nelle nuove tecnologie destinate alla prevenzione degli infortuni. In terzo luogo, una serie di emendamenti è rivolta più generalmente a quell'approccio - che abbiamo considerato doversi privilegiare - per obiettivi. Poco fa il collega Treu dava di questo approccio una versione non corrispondente alla nostra tesi, secondo la quale l'approccio per obiettivi sarebbe in certa misura confliggente con quello per regole. Invece noi riteniamo che l'approccio per regole debba avere il complemento dell'approccio per obiettivi, in modo tale che non si segua la via che questo disegno di legge sembra indicare dell'ulteriore esasperazione degli adempimenti formali, anziché anziché stimolare quanto più la realizzazione di ciò che effettivamente costituisce una prevenzione adeguata rispetto al crearsi dell'evento dannoso. Quindi proponiamo un sistema di monitoraggio presso il CNEL, condiviso dalle parti sociali e dalle istituzioni centrali come da quelle regionali, utile ad orientare le politiche attive rivolte alla salute ed alla sicurezza del lavoro, così come sottolineiamo con forza il ruolo degli enti bilaterali, di quegli organismi che promuovono concordemente le parti sociali e che garantiscono, soprattutto nel tessuto delle imprese diffuse - ove si concentra maggiormente l'infortunio nel lavoro (quindi nell'artigianato, nell'edilizia, nell'agricoltura) organismi bilaterali che dovrebbero garantire semplificazione degli adempimenti attraverso quel controllo sociale che garantiscono. garantiscono. Nel disegno di legge varato dalla Commissione c'è un accenno agli enti bilaterali, frutto proprio della nostra iniziativa emendativa, che però è francamente insufficiente, perché non garantisce alla bilateralità un'adeguata condizione di vantaggio, tale da incentivare l'organizzarsi degli organismi bilaterali. Mi riferisco, ad esempio, alla possibilità di svolgere attività ispettive e di certificare la corrispondenza dei presidi di sicurezza alle disposizioni vigenti. L'ultima parte degli emendamenti riguarda l'apparato sanzionatorio. L'apparato sanzionatorio deve avere caratteristiche di proporzionalità, affinché sia effettivamente utile a prevenire il comportamento delittuoso, la violazione.

gli aspetti più gravi e quelli che invece possono essere frutto di una negligenza, per quanto colpevole, quando arriva poi a prevedere l'interdizione degli amministratori o la sospensione dell'attività dell'impresa, colpisce quei terzi incolpevoli che certamente sono i lavoratori, mette a rischio la stabilità dell'attività produttiva e certamente non scoraggia quegli ambiti di impresa nei quali si concentrano gli infortuni. Mi riferisco a quelle imprese che, muovendosi nel sommerso o a cavallo tra l'attività legale e quella illegale, non hanno certo il timore di sparire per ricomparire poi rapidamente sotto altre forme organizzative. ancora di superare quell'utile alternatività tra l'arresto e l'ammenda che consente la scelta del ravvedimento operoso e quindi della rimozione dei fattori che possono determinare il crearsi del danno per il lavoratore. Il ravvedimento operoso si applica soltanto se c'è la possibilità di sostituire l'arresto con l'ammenda. Invece qui, in alcuni casi, si reintroduce per la prima volta la non alternatività dell'arresto con l'ammenda, eliminando in questo modo la via del ravvedimento operoso che ho sottolineato. Potrei ancora ricordare

e la realizzazione di buone prassi. Cioè, al di là di quanto dispongono in modo cogente le norme, che spesso risalgono addirittura agli anni Cinquanta e che descrivono tecnologie di quel tempo, la possibilità di richiedere all'impresa, sulla base di un'attività ispettiva e di un potere di disposizione conferito agli ispettori, tecnologie più recenti, appunto di quei di quei comportamenti che corrispondono alle buone prassi che sono state monitorate. In tal modo, se l'azienda non adempie, se l'azienda non corrisponde alla disposizione che le è stata rivolta, allora sì che si determina la sanzione. Questo percorso, ancora una volta, corrisponde all'approccio per obiettivi e non solo all'approccio formalistico. Insomma, i nostri emendamenti attraversano questo provvedimento e cercano di ricondurlo ad una logica che voglia davvero creare le condizioni per ricondurre il fenomeno a una dimensione ancora più contenuta

di Governo, tutto formale e formalistico, tutto ispirato ad adempimenti, nel presupposto che l'impresa sia di per sé un luogo pericoloso per il lavoro e per il lavoratore, anzi, come ricordava il collega Ferrara prima,

non corrisponde alle persone che lavorano in carne ed ossa, ai rapporti di produzione quali si determinano effettivamente nella realtà, quella realtà nella quale noi vogliamo intervenire con norme verosimili, per obiettivi verosimili di reale tutela della salute e della sicurezza nel lavoro, secondo obiettivi quantificabili perché la buona politica si deve sempre più misurare con i risultati.

di ritirare gli emendamenti 1.6 e 1.0.2, in qualche modo coperti dall'ordine del giorno

alla tipologia di concentrazione di lavoratrici e lavoratori e alle peculiarità ambientali. È chiaro che gli organici della vigilanza devono essere rapportati a queste condizioni territoriali per poter essere efficaci. Sempre in questo emendamento viene richiamata anche con forza la necessità del principio di cautela rispetto all'esposizione a sostanze tossiche di lavoratrici e lavoratori. L'emendamento 1.1, che è abbastanza articolato, ha però una filosofia e una proposta molto semplice: tende ad allargare su diversi terreni i poteri e le prerogative dei RLS

efficacia, tenuto conto anche dei ricatti e delle debolezze con cui si trovano molte volte ad operare i RLS. Per quanto riguarda l'emendamento 1.2, che va in una direzione completamente opposta

con rapporti di forza molto negativi per le organizzazioni sindacali e per i lavoratori in genere. La mia preoccupazione è rispetto alla valorizzazione di quei tipi di accordi e quindi preferirei affermare la forza della norma.

riferimento ai criteri cui sostanzialmente si ispirano anche i Paesi avanzati - che sono poi i criteri della condivisione e del partenariato

e le difficoltà per l'imprenditore puntino verso un decremento e non verso un incremento. E poi dovremmo che la si smetta anche con il tipo di impostazione secondo cui, per esempio, persino per quanto riguarda la tutela della salute sui luoghi di lavoro bisogna avere particolare riguardo alla differenza di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Perché particolare riguardo? non devono essere sui luoghi di lavoro tutti quanti identici di fronte a misure di prevenzione e di repressione? Che significa particolare riguardo? Cosa significa questa presenza di presunte quote all'interno del mondo del lavoro di lavoratori per i quali bisogna avere particolare riguardo? Mi rendo conto che queste non sono altro che

migranti non si è *à la* *page* sostanzialmente, e non si è promotori di produzione legislativa politicamente corretta. Ma cosa c'entrano queste cose? Stiamo parlando di un disegno di legge, di una legge quadro, di una legge delega la quale deve fare in modo che sia razionalizzato e semplificato tutto il sistema normativo in materia di sicurezza del lavoro. Questi richiami certamente non aiutano anche perché dovete riflettere su quale può essere l'obiettivo anche disarticolatore delle realtà produttive con un tipo di richiamo normativo del genere. Immaginate un richiamo normativo del genere, che lascia ampia discrezionalità giurisdizionale, nelle mani di un magistrato che vuole disarticolare il sistema produttivo; un magistrato con questo tipo d'impostazione non solo può disarticolare, ma anche discriminare tra un'azienda e l'altra. Pertanto, abbiamo presentato questi tre emendamenti per fare in modo che si ritorni alla corretta impostazione di tutta la questione della sicurezza del lavoro: un'impostazione che punta al partenariato, alla cooperazione e che tende

di modifiche di poco conto, ma significative e, mentre nel prosieguo potremo intervenire con dichiarazioni di voto, credo che se il relatore, prima di dare il parere, non intervenga per spiegarci il motivo della proposta, non avremo più la possibilità di averne contezza.

Domando di parlare. PRESIDENTE. Senatore Ferrara, non c'è un obbligo di motivazione del parere, se è per questo. Non apriamo la discussione sul motivo.

Colleghi, vi saranno diverse votazioni: togliete le schede in eccesso, per cortesia.

Presidente, la ringrazio per il controllo posto per posto. Mi pare che questa sia la formula giusta per garantire che tutti votino solo Poi, Presidente, le chiederò qualche volta di fare altrettanto anche con riguardo ai banchi del centro-destra e lei certamente lo farà.

Presidente, voterò a favore di questo emendamento, specialmente visto che, nonostante le richieste, il relatore, che pure ha presentato e dato parere favorevole all'emendamento che in Commissione ha dato luogo alle parole che qui si vogliono emendare, non ha minimamente motivato perché

sono scritte certe parole. Ho chiesto quali differenze ci sono nella tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro tra un lavoratore immigrato e un lavoratore non immigrato.

cosa possibile, data la razionalità con cui agisce il Governo in frequenti occasioni - oppure c'è il trucco: si vuole nascondere qui un ennesimo tentativo di allargare le maglie dell'immigrazione. Non si tratta forse dell'ennesimo tentativo di regalare permessi di soggiorno a lavoratori che, magari, si trovano in ambienti insalubri? Lo chiedo. Mi sembra legittimo pensare che potrebbe trattarsi di questo, visto che il Governo su questo punto sta agendo con un disegno di legge

Dove i lavoratori immigrati hanno una tutela della salute che sia superiore o inferiore o diversa da quella dei lavoratori italiani? Mi piacerebbe davvero saperlo. Si potrebbe citare quel passo di Shakespeare dove il prestatore di soldi ebreo dice: «Forse che se ci pungiamo non proviamo anche noi dolore?». A quanto pare, secondo il Governo ed il relatore,

Presidente, non voglio sostituirmi al relatore, però potrei dare un'interpretazione di natura tecnica che vorrei che l'Aula attentamente considerasse, atteso che di queste cose me ne occupo da tanto tempo. Sarebbe interessante sapere se il relatore abbia mai visto una fabbrica in vita sua. *(Commenti

come potrebbero interpretare la norma gli ispettorati locali e le ASL preposte ai controlli

come minimo, dei lavoratori presenti in fabbrica, con un aggravio enorme di costi burocratici per le aziende. Noi riteniamo che chi viene a lavorare in Italia debba essere tenuto a conoscere la lingua italiana,

manovalanza e di prestazioni d'opera extracomunitaria, rischiamo veramente di costruire una Babele dal punto di vista della documentazione. Rifletterei un attimo sulla questione. Non so se ho rubato il mestiere al nostro muto relatore,

Non riesco a capire cosa c'entri un'attività di tipo professionale con una provenienza di carattere nazionale, a meno che nella testa dei nostri colleghi non vi sia una identificazione per natura,

ad altre, ad esempio forme di tutela speciale che ad altri non vengono assicurate, in nome di un'ideologia o di un concetto di favore verso chi sarebbe in qualche modo penalizzato dalle nostre normative.

quanto dalle sue parti, soprattutto nelle fabbriche dove si sta male, i lavori peggiori li svolgano gli immigrati i quali, essendo spesso meno tutelati degli altri, si trovano nella condizione di subire di più

che oggi le donne e i lavoratori immigrati, sia maschi che femmine, beneficiano di minori tutele oggettive rispetto alla propria salute: lo dicono le statistiche.

che i colleghi della sinistra interpretino la Costituzione in maniera elastica, come il tessuto epiteliale delle gonadi maschili, ma vorrei richiamare l'attenzione del collega

Come fate voi che siete i cultori della Costituzione ad introdurre princìpi che differenziano per provenienza geografica? A noi andrebbe anche bene, perché di cose da dire ne avremmo tante, però tutto ciò mi pare un pochino in contrasto con il vostro abituale modo di ragionare.

garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali». formula, quella originaria del disegno di legge, che non farebbe una piega, perché riconosce un principio elementare, principio dell'uguaglianza, il principio per cui i livelli essenziali in materia di diritti civili e sociali devono essere validi per tutti, senza distinzioni di sesso, razza, religione e via discorrendo. La Commissione ha aggiunto una frase che contraddice in maniera significativa questa regola costituzionale. Non è una regola operativa, parliamo di diritti e non di attuazione dei diritti sul territorio nelle varie realtà locali nelle quali poi si dispiega la tutela del lavoro. La parte aggiunta che si propone di sopprimere

di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati». Ciò significa che, in base a questa aggiunta che proponiamo di togliere, ci sono soggetti che hanno diritti speciali e soggetti che hanno diritti ridotti. Questa formula è assolutamente inaccettabile, poiché - ripeto - mentre nella operatività, nell'attuazione può essere posta una attenzione diversa per situazioni di disagio o di particolare debolezza,

insanabile, per cui vorrei invitare a svolgere una riflessione seria sul punto, che tra l'altro indirizza la delega, che quindi sarà rilevante sul piano

le norme relative alla tutela della salute e sicurezza del lavoratore e della lavoratrice. Non c'è dubbio che differenze antropologiche e fisiologiche determinano - per esempio - la necessità di dispositivi di protezione individuale assolutamente più robusti nel caso del genere femminile, ossia della lavoratrice, e le statistiche relative alle lavoratrici corrispondono effettivamente alla necessità

che gli infortuni sono più presenti fra i lavoratori immigrati - come è stato già detto - in relazione ai *bad jobs* nei quali essi si concentrano, in quanto sono lavori rifiutati molto spesso dai cittadini residenti. In questo caso, però, la statistica non si può in alcun modo risolvere in adempimenti o obblighi maggiori per il datore di lavoro,

L'emendamento 1.41 è davvero rilevante. Tocca un aspetto della complessiva riforma e della produzione del Testo unico, che poi tornerà in altri emendamenti. Infatti, qui si propone che si affermi - quale criterio ispiratore della della intera disciplina - la commisurazione degli adempimenti alle caratteristiche settoriali e dimensionale delle aziende. Il problema si pone perché tutto il sedimento normativo, che qui dovrà essere riunito, semplificato ed anche in parte sottoposto a novazione, è essenzialmente costruito sull'impresa di grandi dimensioni, strutturata, organizzata, alla quale si chiedono adempimenti sostenibili da questa dimensione d'impresa. Ma proprio per la volontà di rendere le disposizioni più effettive, rispetto al grado di ineffettività che largamente riscontriamo, in particolare nelle piccole imprese, è importante che vi sia da parte del legislatore la capacità di adattare molte disposizioni alla dimensione aziendale, alle caratteristiche quindi anche settoriali dell'impresa; che cioè la disciplina si articoli quanto più in modo da essere, come diciamo sempre, effettiva, in modo da avere ragionevolmente una prospettiva di effettiva applicazione. Per questa ragione, l'emendamento 1.41 va sostenuto, così come sosterremo altri emendamenti nostri e di altri colleghi che sempre si riconducono a questo fondamentale obiettivo: avere disposizioni che si articolano,

n. 626 è intervenuto nella nostra legislazione con gravi conseguenze dal punto di vista organizzativo ed anche economico, sopratutto sul tessuto delle piccole e medie aziende, ormai da quasi dieci anni perché, di fatto, comincia ad essere applicato intorno al 1996. Vi è un dato curioso, nel modo più assoluto, in tutto ciò:

legati soprattutto alla modernizzazione dei cicli tecnologici. Oggi le macchine sono quasi tutte automatiche, quindi è evidente che chi lavora sulle macchine automatiche si fa meno male di chi lavora sulle macchine manuali. Se andiamo a vedere questa curva, ci rendiamo conto che essa non è stata modificata in nulla dall'intervento del decreto legislativo n. 626. Cioè, l'incidentalità e la mortalità in Italia nelle aziende manifatturiere ha continuato a diminuire esattamente con lo stesso *trend* che aveva prima che venisse introdotto il decreto n. 626. Questo ci dovrebbe far riflettere.

adempimenti che poi, fuori di qui, non qui dentro, le piccole e medie aziende dovranno tradurre in adempimenti concreti e che rischiano di rimanere soltanto sulla Torno rapidamente sulla questione dei lavoratori e delle lavoratrici extracomunitari. È vero che, abituati a noi stessi, forse diamo scarsa fiducia al legislatore, forse questo è il dato; decreto n. 626 distingue chiaramente le donne dagli uomini, è del tutto ovvio. Pensiamo soltanto alle norme per il sollevamento dei pesi;

che verrà cassata dalla Costituzione, perché il diritto alla salute e il diritto alla sicurezza sono diritti universali che non possono essere rescissi e scissi in funzione del genere e della provenienza. Quindi, sarà una norma che sicuramente cadrà sotto la mannaia della Corte.

1.30, che fa riferimento al comma 2 dell'articolo 1, laddove, all'inizio, si dice che i decreti di cui al comma 1, cioè il decreto

l'applicazione della normativa in materia di salute sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio: ebbene, a tale proposito non è stata accettata la correzione che ciò fosse fatto con un elemento salvifico rispetto ai principi della commisurazione degli adempimenti di funzione. C'è ancora la possibilità di dare la giusta correzione alla proposta che proviene dalla Commissione, quella di aggiungere, dopo le parole «tipologie di rischio», soltanto tre parole che avrebbero il significato di ricondurre la disposizione all'interno, se non propriamente nel perimetro esatto, così come richiesto dall'emendamento 1.41, o almeno in un perimetro un po' più allargato, ma comunque più

un sedimento normativo che nella raccolta di tutto ciò che è stato fatto, detto e scritto, degli indirizzi che sono stati tracciati, ha come punto ultimo il raggiungimento di obiettivi che in primo luogo cercano di ricondurre i grandi insediamenti al rispetto delle normative e quindi, in tal senso, a far sì che l'applicazione determini una conseguenza culturale e un rispetto delle normative: in una parola, una linearità, dalle aziende più grandi a quelle più piccole. Ma cosa consegue da un'applicazione di una delega così estesa?

rinuncia da parte delle piccole aziende al conseguimento dei perimetri di sicurezza e quindi, a questo punto, un danno economico, che è il motivo per cui in Commissione bilancio ci siamo battuti affinché la delega non fosse generica e indicasse

proiettata soltanto nei decreti successivi. In questo modo, il raggiungimento degli obiettivi potrebbe essere svilito, sminuito, non realizzato e in questo senso la correzione richiesta

e sicurezza sul lavoro a tutti i lavori. Questo era un obiettivo già presente nella legge Biagi, che ha esteso le tutele fondamentali in materia di tutela e sicurezza sul lavoro

prevedeva di estendere - per la prima volta, peraltro, nel nostro ordinamento - ai lavoratori autonomi alcune misure relative alla loro salute e sicurezza, e sicurezza, mentre i loro dipendenti sono ovviamente già tutelati dalle disposizioni vigenti. Vorrei ricordare, inoltre, che la Commissione europea non ha raggiunto

sanitario. La premessa per un emendamento di questo tipo, che successivamente esamineremo, è di eliminare il riferimento ai lavoratori autonomi, perché per essi deve valere una disciplina speciale che, come ho detto, li consideri destinatari, oggi e non ieri, delle norme che mirano a proteggere la tutela e la sicurezza sul lavoro, ma in una dimensione del tutto speciale, come del

ieri sera, a conclusione della seduta - e quindi successivamente alla comunicazione dell'ordine del giorno di oggi - è stata presentata dal prescritto numero di senatori la richiesta di rimessione all'Assemblea del parere della 1a Commissione permanente sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge sulla liberalizzazione dei mercati energetici. Ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, la deliberazione dell'Assemblea deve avvenire entro cinque giorni. Il Senato è pertanto convocato lunedì 25 giugno, alle ore 18, per la predetta deliberazione.

*(Ulivo)*. Signor Presidente, nel dare appuntamento ai colleghi per lunedì alle ore 18, volevo chiederle una cortesia: se può interporre i suoi buoni uffici affinché la prossima volta, verificandosi le stesse circostanze, sia possibile procedere ad esprimere il voto sui presupposti nella giornata di giovedì, anziché nella giornata di lunedì. Mi pare utile per il buon andamento dei nostri lavori. Capisco che, forse, questa volta non si è potuto fare, ma in futuro

e inserisce; questo perché si legge: "sottopone (...) al voto dell'Assemblea", e non si parla di inserimento all'ordine del giorno. Quindi, avrei dato una lettura come la sua. Non essendovi oggi il Presidente in sede, si è preferita questa strada che mi sembra più elegante e accettabile.